La seduta è ripresa. Invito i colleghi a ritirare la tessera, a prendere posto e ad inserirla nell'apposita fessura in modo da poter procedere alla

parere favorevole.

nella coscienza dei consumatori è iniziato un percorso che porta sempre più ad affermare l'importanza delle informazioni contenute nelle etichette. Basti pensare che, secondo una ricerca dell'ISPO, otto italiani su dieci considerano necessario che sia indicato in etichetta il luogo di origine della materia prima. Ebbene, l'Europa ci ha detto che ciò non è possibile, perché il Regolamento delle dogane prevede solamente la necessità di indicare il Paese di produzione,

si rendeva necessaria da parte del Governo una risposta senz'altro positiva alle mozioni presentate, in particolare

Il Governo esprimeva pertanto parere favorevole. In quest'Aula abbiamo votato una mozione trasversale,

Quindi, delle due l'una: o il Governo in quel momento ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e si è impegnato a non toccare

Petris, che la mozione che noi abbiamo condiviso e votato insieme a lei prevedeva di non toccare in alcun modo la legge del 2004. Se vuole, le faccio vedere gli atti.

ovvio che l'Europa ci ha minacciato di infrazione, ma è anche evidente che non è detto che dobbiamo seguire sempre pedissequamente quello che ci dice l'Europa

Grazie, Presidente.

di abrogare la legge n. 204 che noi invece chiediamo di difendere. Pertanto, senatore Polledri, nel testo proposto dalla Commissione, proprio quell'articolo 7 del testo iniziale del Governo è soppresso

Presidente, la senatrice De Petris ha già chiarito bene il problema: l'articolo 7 del testo del Governo è stato soppresso in Commissione, in conformità con quanto votato e approvato in quest'Aula relativamente alla

senatore Polledri, *nulla quaestio*, nel senso che proprio come aveva deliberato quest'Aula, l'articolo 7, proposto dal Governo, è stato soppresso dalla Commissione e quindi la legge n. 204 del 2004, che norma

Signor Presidente, confermo quanto è stato appena asserito dai colleghi. Peraltro la preoccupazione del senatore Polledri non è campata in aria,

produce norme di legge in contrasto con questi princìpi che invece ci vedono tutti quanti solidali. Mi pare che l'avvertimento preoccupato del senatore Polledri possa essere in qualche modo recepito e

solo una settimana fa vi è stata una grossa manifestazione organizzata dalla Coldiretti che ha portato 150.000 agricoltori in piazza a protestare doverosamente contro il ministro De Castro e soprattutto contro il Governo Prodi. quindi che questa buona volontà è stata sicuramente agevolata anche da una forte manifestazione di piazza, voluta dai nostri contadini, categoria della quale mi onoro di far parte.

Sarebbe assolutamente sbagliato modificare questo tema, visto che poi su di esso si basano anche il prezzo al consumo e quindi i diritti dei consumatori. Colgo l'occasione, se mi è consentito, per elevare una lamentela: senza nulla togliere alla valentia del Sottosegretario alla giustizia, su questi temi deve rispondere la signora ministro Bonino, altrimenti non ha senso. Una competenza per materia deve essere rispettata, se la signora ministro Bonino non è in Aula, sospendiamo la seduta fin quando non arriva, ma avere un parere come è accaduto poc'anzi, in cui il relatore si rimette al Governo, il Governo si rimette all'Aula e l'Aula non si sa a chi si rimetta, francamente mi sembrerebbe fuori luogo.

L'articolo introdotto in Commissione, se approvato, creerà un grave danno per quegli impianti che sono già stati autorizzati, ma che ancora non sono stati costruiti. In tutta Italia sono soltanto sei gli impianti di questo tipo: quattro in Sicilia, uno, mi sembra, in Calabria ed uno sicuramente a Torino.

se non c'è accordo di concerto tra il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico non esiste in questo articolo la possibilità di intervenire, quindi si può restare per anni a discutere se riconoscere o meno la deroga sul provvedimento. Credo che tutto questo non sia assolutamente accettabile, a meno che

si rischia quello che sta accadendo ormai da tanto tempo in Campania, visto che i due impianti della Campania non sono stati costruiti: uno è ora in fase di costruzione; l'altro deve ancora partire. È bene che coloro

*(UDC)*. Intervengo per appoggiare, signor Presidente, senatori colleghi, le argomentazioni svolte dal presidente Matteoli. Nel caso specifico della Regione siciliana, si tratta anche di dar corso ad un'intesa realizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il Presidente della Regione. L'eventuale approvazione del testo, così com'è formulato, impedirebbe in Sicilia la realizzazione degli impianti già coperti da un impegno finanziario assicurato dal sistema bancario.

per la pressante posizione radicale, probabilmente di qualche parte della maggioranza. Signor Presidente, non per essere ripetitivo rispetto a quanto è già stato rappresentato dai colleghi che mi hanno preceduto - mi riferisco ai senatori Vegas e Matteoli ma con l'emendamento approvato in Commissione sul disegno di legge comunitaria n. 1448/A, all'articolo 8 si è inserita la modifica del comma 1117 (articolo 1 della legge finanziaria Tale comma disponeva che i finanziamenti e gli incentivi pubblici finalizzati alla promozione di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica siano concessi anche per gli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione. Il comma 1118 stabiliva poi che il Ministro dello sviluppo economico provveda, con propri decreti, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento, in deroga al diritto agli incentivi, a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio. Il nuovo articolo 8 sullo stampato n. 1448/A prevede una modifica del comma 1117, nel senso di concedere finanziamenti ed incentivi ai soli impianti realizzati ed operativi. Alla luce di tale nuova disposizione, rimarrebbe escluso ad esempio l'inceneritore di Acerra, un impianto in fase di completamento, rispetto al quale sono già stati spesi 600 miliardi di vecchie lire e ora, per pochi miliardi, rischiamo di non completare l'opera. La disposizione in questione era già stata oggetto di un tentativo di inserimento nella legge di recepimento di direttive comunitarie approvate dal Senato nel febbraio scorso. In quella sede i Capigruppo di maggioranza erano riusciti a trovare un accordo consistente nell'esclusione di tale disposizione da quel disegno di legge, poiché controversa e meritevole di approfondimento in autonomo disegno di legge, peraltro già presentato in corrispondenza al disegno di assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 10a e 13a, il cui esame non è ancora iniziato. Alla luce del suddetto quadro, vorrei chiedere al relatore, ai colleghi della maggioranza e al Governo se l'approvazione di tale disposizione non risulti fortemente in contrasto con l'esigenza impellente di risolvere l'emergenza rifiuti in Campania, che ci ha portato all'approvazione, qualche mese fa, di un provvedimento, il famoso decreto Bertolaso.

Signor Presidente, credo che ci sono almeno due Regioni italiane (probabilmente anche altre, ma due le conosco bene) che da questa norma vengono messe in una situazione di grandissima difficoltà:

di non bloccare il termovalorizzatore che finalmente si è riusciti a costruire e credo che esattamente la stessa situazione vi sia nella Regione Sicilia, con quattro termovalorizzatori, e in diverse altre Regioni (io conosco queste due), che sono in una situazione analoga. Si tratta di impegni di spesa presi. Si tratta di Regioni che rischiano di spendere una montagna di denaro per nulla. Si tratta di impegni che possono essere fatti valere in tribunale da chi può citare, perché sono stati dati affidamenti che non si è in grado di mantenere. Questa norma è l'espressione plateale di un'ideologia che vuole imporsi piegando a forza la realtà. Almeno le situazioni pregresse andavano salvaguardate. Invito pertanto tutti i senatori a votare contro questa norma di legge. Devo poi dire, signor Presidente, passando all'ordine dei lavori,

nome abbiamo dato al Ministro per le politiche europee forti poteri di coordinamento. Egli è il presidente di una specie di CIPE, di un Consiglio dei ministri *ad* *hoc* per le questioni comunitarie, ed è responsabile per la politica comunitaria. Non è pensabile che l'approvazione della legge comunitaria venga ridotta ad una specie di adempimento burocratico, ad un atto dovuto, senza che possano essere messi effettivamente in discussione i grandi orientamenti della politica europea, che sono i grandi orientamenti della politica nazionale. alla questione delle pensioni: esiste un tema più europeo di questo? È sulla questione delle pensioni che rischiamo di essere cacciati dall'Unione Europea se non manterremo gli impegni presi, e così via

se risultasse che il Ministro è occupato a spiegare la sua linea politica ai giornali o a discuterla all'interno della coalizione, quando rifiuta di venire ad esporla in Parlamento Signor Presidente, la prego di farsi interprete della domanda dell'Assemblea di avere qui presente il Ministro e non un Ministro dimezzato, ma un Ministro che risponda a questioni politiche, con una chiara, precisa e convincente linea politica. Se non è in grado di farlo perché la sua maggioranza non lo appoggia, rinviamo, si dimetta, chieda che si tenga il dibattito dopo che avrà chiarito i problemi di linea politica europea all'interno del Governo. Oppure venga e chieda i nostri voti e le assicuro che saremo felici di darglieli per cose utili all'Italia e per una vera ed autentica politica europea.

non ci sono solo quelle due Regioni, c'è anche la Lombardia, per cui l'appello lo rivolgiamo anche ai parlamentari lombardi. Vede, Presidente, abbiamo già detto che sul CIP6 in passato si è consumato denaro e anche oggi il CIP6 costa alle tasche dei contribuenti circa 5 miliardi di euro.

perché abbiamo considerato assimilati alle fonti rinnovabili alcuni derivati del petrolio. Abbiamo considerato assimilato alle rinnovabili tutto quello che non era rinnovabile.

le immondizie: vanno in piazza e tutte le volte facciamo un decreto. Colleghi, non è che le immondizie si fanno sparire - «abracadabra» - con un decreto. Per le immondizie o si trova un posto dove buttarle o si bruciano; non potete farle sparire per decreto.

Vorrei ricordare che il testo dell'emendamento, così come riscritto all'interno della legge comunitaria, è lo stesso che, soltanto per un mero errore di trascrizione, era già previsto nella finanziaria 2007, così come il ministro Chiti comunicò all'Aula, chiedendone un aggiustamento formale, il senatore Matteoli sollevò il problema che si trattava di una differenza tra impianti realizzati e impianti autorizzati, per cui abbiamo accettato quella soluzione e siamo andati avanti. Vorrei precisare che quando si parla di CIP6

Ricordo ancora al senatore Buttiglione che l'onorevole Tabacci ha definito quella dei CIP6 una truffa legalizzata all'interno del panorama politico del nostro Paese. Mi appello a quanti accusano la mia parte politica di essere poco attenta alle riforme, alla concorrenza e al mercato: è una norma di libero mercato consentire a chi in Italia intende costruire ed utilizzare impianti per l'incenerimento dei rifiuti, farlo come in Francia, in Germania, in Inghilterra e in Austria, dove

Esistono 20 richieste di autorizzazione rispetto alle quali, caso per caso, si deciderà la deroga, ma si tratta, appunto, di un'azione successiva. Non possiamo continuare a tenere in vita una

per metterli in discussione con una norma che facciamo oggi dopo dieci anni da una gara di appalto. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di quelle autorizzazioni presentate all'ultimo minuto o per le quali è addirittura in corso un *iter* autorizzatorio non ancora completato. Si tratta di una norma del tutto

mantenere questa anomalia tutta italiana. Questo vogliamo fare con la norma. Vorrei ricordare ai colleghi della maggioranza che su questo argomento c'è stato un impegno. Anch'io aspetto che arrivi la signora ministro

noi. Lo dobbiamo ricordare per dovere e per la stessa tutela dei consumatori. Molti calciatori sono stati pagati con queste risorse, ricordiamocelo sempre. È ovvio che da questo punto di vista dobbiamo rientrare nelle regole; abbiamo fatto una parte del cammino, poi con la modifica

che si prevedesse la possibilità di una deroga in capo al Ministro dell'economia, di concerto ovviamente con il Ministero dell'ambiente, che è l'altro titolare. Quindi, non ci sono accanimenti e non inventiamoci crisi napoletane, perché la crisi della Campania è la testimonianza del fatto che avere l'idea di gestire i rifiuti puntando soltanto sui termovalorizzatori produce quello che produce. Vorrei inoltre ricordare (lei dovrebbe conoscerlo altrettanto bene, caro senatore Matteoli) il consorzio Gaia

sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi», perché non aggiungere (senza ricorrere alle deroghe, perché sappiamo che già Pecorario Scanio non vorrà autorizzare questa deroga)

sia pure telegraficamente (avendone già enunciato sostanzialmente tutte le ragioni di merito il presidente Matteoli, riprese poi da altri colleghi intervenuti), sull'emendamento 8.103, che si pone in una linea gradata e subordinata rispetto a quelli soppressivi, essendo sostitutivo dell'articolo ed avendo lo scopo di far salvi i diritti quesiti di coloro che, ottenuti i relativi decreti di autorizzazione, avendo avviato le conseguenti procedure avendo ottenuto finanziamenti da istituti di credito, abbiano già dato inizio alla realizzazione degli impianti. In questa breve illustrazione delle motivazioni dell'emendamento, che - ripeto - si pone in posizione subordinata e gradata rispetto a quelli soppressivi... Presidente, lei sa che normalmente sono scevro da qualunque notazione polemica, ma è evidente che anche i mezzi dialettici, dei quali pur dispongo, di fronte al brusìo dell'Aula di fatto soccombono impedendomi

invenzioni legislative, ha richiamato precise leggi dello Stato all'epoca vigenti e tali, quindi, in quanto leggi dello Stato, da determinare, in favore di coloro che di quelle leggi si avvalevano, dei diritti quesiti. quesiti. È un punto fondamentale sul quale mi pare non sia stata fatta assolutamente chiarezza. Non voglio riprendere argomentazioni già ampiamente illustrate dai colleghi, che attengono a tutte le conseguenze di merito che deriverebbero dall'approvazione dell'articolo 8, così come impropriamente formulato. Vorrei però che si riflettesse attentamente su un aspetto: aspetto: parliamo di sei-sette impianti in corso d'opera, attualmente in fase di realizzazione perché, vigente una legge dello Stato, si è dato corso a ciò che quella stessa legge prevedeva, determinando evidentemente in coloro che se ne sono avvalsi dei diritti che devono comunque essere rispettati, salvo voler introdurre un inammissibile principio di retroattività sfavorevole della legge, il che è assolutamente impensabile ed inammissibile, a prescindere da tutte le conseguenze che ciò fatalmente determinerebbe per lo Stato a fronte delle azioni che legittimamente verrebbero proposte contro lo Stato medesimo. Vi è di più, come opportunamente il presidente Matteoli, con garbo ma con fermezza, tra le righe ha fatto trapelare, onorevoli colleghi. Perché il meccanismo della deroga, quando ci troviamo di fronte a sei impianti che sono in punto di fatto e di diritto esattamente nelle stesse condizioni? Perché si pensa di poter determinare una disparità di trattamento fra sei situazioni assolutamente omologhe in punto di fatto e di diritto, al di là di tutte le disastrose conseguenze di merito che bene sono già state illustrate? È assolutamente incomprensibile. Qui di truffe non ve n'è alcuna. Semmai - ed è questa la vera grande preoccupazione che traspare leggendo l'articolo perché non si vuole prendere atto che ci troviamo di fronte a sei iniziative in avanzatissima fase di realizzazione, avviate in base ad una legge vigente dello Stato, con significative esposizioni di coloro che di quella legge si sono - ripeto - legittimamente avvalsi e dei quali - non si sa attraverso quale percorso - si arriva ad ipotizzare una potenziale disparità di trattamento. Badate bene, l'emendamento,

approvassimo il testo proposto all'Aula dal Governo e dalla maggioranza, esporremmo consapevolmente, deliberatamente e ingiustificatamente lo Stato italiano ad una serie di gravose ed onerosissime controversie che dovremmo dare di per sé perdute in partenza, con tutti i danni per l'Erario che ciò comporterebbe. Signor Presidente, colleghi, nei giorni scorsi abbiamo tutti ricevuto una lettera firmata dai Radicali italiani, la formazione politica alla quale appartiene il ministro Bonino, cui ci si informa che «Il Comitato nazionale dei Radicali italiani ha deliberato un'immediata mobilitazione di opinione pubblica e istituzionale perché vi sia una grande riforma parlamentare e politica: immediatamente sia resa pubblica tutta la documentazione sui comportamenti istituzionali di tutti i deputati e senatori nell'esercizio della loro funzione, nelle loro attività e in attività parlamentari». Ora, la formazione politica del ministro Bonino ci invita a denunciare il fatto che lo stesso Ministro Bonino non sta rispettando il suo dovere politico-parlamentare e istituzionale di essere presente nell'unica occasione in cui le è fatto obbligo di essere presente in Parlamento.

Si sospende dunque la seduta fino a quando il Ministro non arriva e non rispetta, se non la Costituzione, almeno i deliberati del suo partito.

faccio appello ai colleghi eletti in quella Regione - non esiste un problema rifiuti come esiste, purtroppo, a Napoli e in Campania. In Calabria funziona da anni un termovalorizzatore costruito da un'impresa privata socia della Banca Intesa, primo gruppo bancario d'Italia. Nella stessa Regione, proprio perché il termovalorizzatore funziona e gli utenti sono assai contenti del servizio (del resto non si trovano rifiuti per le strade), da un anno e mezzo è stata avviata la costruzione di un nuovo termovalorizzatore, sempre a Gioia Tauro. A seguito delle iniziative del Governo, le società bancarie finanziatrici di quel termovalorizzatore hanno comunicato alla società promotrice l'intenzione di revocare i fidi.

per quale motivo non dovrebbe essere possibile da parte di osservatori stranieri ironizzare sulla realtà italiana, dove uno Stato fa riferimento a Berlusconi ed un altro fa riferimento a Prodi. Infatti, un rappresentante del Governo firma un contratto mentre altri avocano a sè un diritto,

che attribuire un improprio diritto di concessione e di veto su misure già approvate. Anche a parer mio la norma deve essere necessariamente modificata, non già per aprire varchi a future iniziative che non si sa bene

Signor Presidente, nell'esprimere il mio rammarico per l'assenza del Ministro, intendo intervenire - come hanno già fatto altri colleghi dello schieramento di opposizione

mentre le deroghe di cui si è parlato (e quindi per situazioni future) dovrebbero prevedere il sostegno di questi impianti, si nega il sostegno degli impianti che hanno la stessa finalità e per di più

si dice che non si concedono più quei sussidi e quelle forme di contribuzione proprie del CIP6,

Grazie, si ledono gravemente i diritti di sei o sette imprenditori che con il *project* *financing* hanno in atto iniziative imprenditoriali che non hanno ancora portato al funzionamento dell'impianto, che però è già stato autorizzato. Si ledono gravemente sacrosanti

artato, la legge comunitaria per introdurre una supposizione che non c'entra nulla con la medesima. Infatti, non è assolutamente vero che il finanziamento di questi sei o sette impianti va a vantaggio delle fonti rinnovabili.

elemento veramente vergognoso. L'Unione Europea non fa altro che raccomandare procedure

che ha presentato un proprio decreto, venga in Aula e non sia consapevole che il Presidente del Consiglio abbia già concertato con il Presidente della Regione siciliana al fine di realizzare i termovalorizzatori in Sicilia. È incredibile che non ci sia la sensibilità politica per poter apprezzare come questo Governo sia in balìa di un mare tempestoso e non sappia dove deve andare.

in particolare, dovrebbe sapere quanto costa, visto che il problema che interessa i colleghi intervenuti è quello di garantire, possibilmente, gli interessi legittimi dell'imprenditore che ha fatto degli investimenti. Mi chiedo se qualcuno si sia posto l'interrogativo quali sono i veri interessi da tutelare, se non quelli del cittadino, che ad oggi, caro collega parlamentare siciliano eletto nella provincia di Palermo, paga l'immondizia 700 lire al chilo per farla trasferire nella discarica di Bellolampo. si vuole far diventare la Sicilia come la regione Campania, si vuole consentire la politica disastrosa che il centro-sinistra sta realizzando con le frange estreme della sinistra, che immediatamente dopo l'elezione del presidente Prodi a Presidente del Consiglio, hanno detto che non si debbono realizzare i termovalorizzatori, che non si deve realizzare la grande opera

da realizzare, ad un certo punto, si alza il ditino, mentre il Presidente del Consiglio cerca il concerto con il Presidente della Regione, ecco che allora un Governo assente non sente il dovere d'intervenire

voi che andate alla ricerca della qualità della politica, della trasparenza della politica, cosa significa cercare di concertare, di perdere tempo sul piano delle deroghe. Questo significa non voler rispondere alle esigenze del territorio, prendere in giro la gente, questo significa non creare elementi di produttività e di evoluzione di una Regione o di Regioni che hanno necessità di rispondere all'esigenza del territorio. La Sicilia, come le altre Regioni, non può diventare il letamaio della nostra nazione, la Sicilia vuole difendersi e tutelarsi e non vuole essere tutelata da un Governo che tratta con il Governo siciliano per cercare di prendere respiro, sperando di potere avere qualche consenso dai centristi all'interno del Parlamento e poi consente ai propri uomini di presentare un emendamento orientato in senso opposto. Caro presidente Sodano,

vi dovete confrontare con quello che ad oggi è realizzato, voi non potete bloccare il gioco in corso, con le carte date, non potete cambiare le carte in gioco, perché non è corretto, e perché soprattutto mortifica un regolamento. La verità, la vera verità è che voi volete comunistizzare questo nostro Paese e lo volete comunistizzare perché non volete rispettare le regole e le regole sono quelle che noi ci siamo dati, le regole sono quelle che il Parlamento si è dato. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP).* Nel corso di un gioco, le regole valgono per tutti, e quando sono scritte il gioco è fatto, *rien ne va plus*! Ecco per quale motivo chiediamo la soppressione di questo articolo, perché è un obbrobrio ed una mortificazione per la politica e per le regole che valgono per la democrazia e per la garanzia della libertà in questa Nazione.

Presidente, faccio mia l'osservazione del collega Possa, che credo non si possa smentire, a meno che non lo facciano in Aula il relatore o il Governo, che vedo comunque rappresentato da un Ministro che non mi sembra competente nella materia comunitaria. Faccio mia quella dichiarazione in forza della quale l'aggancio alla normativa comunitaria è strumentale per consentire l'ingresso di questa norma nel testo del disegno di legge. Se così fosse,

un chiarimento su che cosa stiamo votando, perché a me sembra chiaro che il testo dell'articolo 8 parli di soli impianti realizzati ed operativi. Se il relatore non mi ascolta, è inutile, Presidente. Se il relatore non ascolta, non posso parlare.

a me sembra che il testo della norma sia chiaro: si parla degli impianti realizzati ed operativi. Poiché i colleghi della maggioranza, il senatore Sodano e la senatrice De Petris in particolare, hanno accennato ad ipotesi diverse da quella prevista dalla norma, cioè che si possa trattare di impianti solo finanziati o in corso di realizzazione, anche se mi sembra chiara la norma, vorrei chiedere al relatore e al Governo quando ci sarà e sarà in grado di esprimersi se essa vuole riferirsi solo agli impianti operativi, che significa gli impianti che già sono funzionanti, e quelli che fossero ultimati ma non funzionanti rientrerebbero invece nella deroga. Questa sarebbe veramente la conseguenza più aberrante della norma introdotta dalla Commissione. Vi chiedo una conferma perché a me sembra che le parole dei senatori Sodano e De Petris vadano in una direzione fuorviante rispetto al testo dell'articolo in esame.

in quanto si tratta di tre emendamenti che combattono l'allevamento degli animali da pelliccia in gabbia, già proibito da questo Parlamento con un voto nel mese di febbraio, più volte proibito dal Parlamento europeo. Il mio voto, quindi, sarà a favore di questi tre emendamenti.

all'equilibrio raggiunto con l'emendamento proposto dalla Commissione, che rappresentava una sintesi rispetto a diverse esigenze. Questo equilibrio viene ad essere ora rotto, non si capisce per quale ragione, senza valutarne gli effetti in maniera adeguata; effetti che colpiscono i nostri allevamenti e determinano forti conseguenze sul piano economico ed occupazionale. Vorrei richiamare l'attenzione dei presentatori sul fatto che in una economia globalizzata è facile superare gli ostacoli ed anche andare in Cina a realizzare allevamenti che non hanno nessuna regola e nessun rispetto; rispetto che noi cerchiamo di realizzare attraverso un equilibrio tra normativa nazionale e raccomandazioni comunitarie. Per queste ragioni, Presidente, invito fortemente i presentatori a rispettare la pronuncia della Commissione affari comunitari, ribadendo la necessità di evitare danni rispetto ad un settore fortemente già colpito e ridimensionato e non deve essere ulteriormente penalizzato. [SCARPA BUORA *(FI)*. Signor Presidente, vorrei ribadire, in modo assolutamente succinto, il concetto appena esposto dal collega Eufemi. Veda, Presidente, vedete colleghi, ad ognuno di noi sta a cuore il benessere degli animali. Negli anni in cui mi è capitato di occuparmi di allevamento a Bruxelles, molto spesso si andava a ragionare sul benessere degli animali e giustamente: una sensibilità che gli agricoltori e gli allevatori - in questo caso gli allevatori di animali da pelliccia - hanno. Credo però che ogni tanto occorrerebbe anche occuparci del benessere degli allevatori. Non possiamo mettere in campo delle norme che finiscono per determinare la chiusura di impianti produttivi che sono stati realizzati e che hanno richiesto impegni finanziari notevoli, nei quali sono impiegate migliaia di persone, a meno che non si voglia invece utilizzare strumenti che purtroppo in passato, e qualche volta anche adesso, sono stati utilizzati dai cosiddetti animalisti. Mi riferisco a quei signori che vanno di notte negli allevamenti di visoni e lì liberano, esponendoli a morte certa, o a coloro che vanno a liberare le lontre, che poi infestano il nostro territorio, mettendo anche a rischio la salute e la sicurezza dei nostri ragazzi e di ognuno di noi. cerchiamo di non esagerare: il benessere degli animali è un valore importante che credo ci accomuna tutti, però occupiamoci una volta tanto anche del benessere dei nostri allevatori e dei nostri allevamenti. pertanto i cari colleghi che, con spirito particolarmente umanitario, hanno presentato questi emendamenti a valutare con attenzione l'opportunità di ritirarli.

Presidente, sono sulla stessa linea del collega Santini, perché penso che questo genere di allevamenti che esiste in Italia debba essere riconvertito. Così come chiediamo la riconversione dei campi di papaveri in Afghanistan, così dobbiamo chiedere la riconversione di qualcosa ormai superato nel tempo e nello spazio come l'allevamento di questi animali, semplicemente

belli o significativi ma che non implicano allevamento e l'uccisione di animali. Bisognerebbe andarli a valutare uno dopo l'altro. In molti casi i servizi televisivi hanno riportato

stiamo parlando finalmente di un sistema di certificazione per il legname per evitare il commercio illegale di questo prodotto. Infatti, è inutile continuare a parlare a parlare di cambiamenti climatici, se poi non mettiamo in atto una serie di strumenti concreti volti ad impedire, ad esempio, la deforestazione di una serie di aree importanti proprio ai fini del clima.

del Parlamento per quanto riguarda la giustizia? Mi domando come si possa delegare il Governo ad elaborare sanzioni così importanti senza che si rispetti questa riserva di legge.

*(UDC)*. Signor Presidente, arriva in questo momento la dolorosa notizia della scomparsa del professor Antonio la Pergola essere stato Presidente della Corte costituzionale, è stato un grande Ministro per le politiche comunitarie e autore della «legge La Pergola» che ha regolato la partecipazione dell'Italia alle istituzioni comunitarie fino ad un paio di anni fa. Credo che tutta l'Aula abbia motivo di meditare con riconoscenza sulla figura di questo grande studioso e grande gentiluomo che ha rappresentato l'Italia anche presso la Corte di Giustizia europea, sempre con straordinaria straordinaria dignità; uomo di studi severi, di grande intelligenza e di straordinaria umanità.

voto sarà sicuramente contrario. Vorrei comunque chiedere alla Presidenza se può essere ammissibile un articolo introdotto dalla Commissione che delega il Governo in materia di sanzioni, cioè in materia penale.

approvano articoli che vengono inseriti, infarcendo provvedimenti di iniziativa governativa o parlamentare, che avevano tutt'altra impostazione.

si possa giustificare dal punto di vista della sorpresa, debba fare una riflessione prima di mettere in votazione un provvedimento con una fortissima lesione costituzionale di questo tipo che, ripeto, essendo stata introdotta in Commissione, non è passata al vaglio della 1a Commissione nella fase dell'esame iniziale del provvedimento, così come vuole il nostro Regolamento e la nostra prassi

che siano informate preventivamente le autorità locali, ma ciò significa che in Italia non si riuscirà a trasportare più nulla e si bloccherà tutto. Mi sembra una cosa assolutamente

Senatore Vegas, vuol dare una mano al Governo? VEGAS *(FI)*. Signor Presidente, mi permetto di ricordare al Governo che questo emendamento mira a ripristinare una prima parte del testo governativo relativo agli IAS (i sistemi contabili internazionali per le imprese), e mi sembra che il Ministero dell'economia

Signor Presidente, il mio Gruppo, da questo momento in poi, si trova in forte imbarazzo, perché stiamo affrontando una legge rilevante, come la legge comunitaria

in cui il relatore si è rimesso al Governo, ma comprendo le difficoltà del sottosegretario Scotti, così volenteroso e attento. Abbiamo una certa difficoltà a votare senza conoscere esattamente qual è la posizione del Governo su punti così delicati. quindi sapere se la Presidenza si è attivata per chiedere al Ministro competente di essere presente e quali risposte si siano ottenute al riguardo, riservandoci di valutare la nostra partecipazione alle votazioni successive sulla base di tali riscontri.

si potrebbe accantonare questo articolo e proseguire con i nostri lavori. Signor Presidente, capisco lo sforzo fatto dal collega Boccia, che mi ha preceduto, che pensa di poter accantonare questo emendamento.

Signor Presidente, mi giunge notizia che il ministro Bonino, il quale evidentemente ha cose più importanti da fare che venire a questa seduta del Senato, trova però almeno il tempo - e lo ringrazio - di incaricare il suo portavoce, il suo addetto stampa di comunicare che è impegnata a presiedere una riunione di esperti Italia-Qatar. Ora, con tutto il rispetto per un importante, anche se piccolo, Stato (il Qatar, per chi non lo sapesse, è uno Stato proprio piccolino che si trova tra gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita), l'Arabia Saudita), vorrei ricordare che un Ministro è, prima di tutto, responsabile verso il Parlamento; è Ministro perché ha la responsabilità del Parlamento nel formulare la sua agenda. Signor Presidente, sono stato Ministro anch'io e ricordo molto bene - ne chiedo conferma a tutti coloro che hanno avuto responsabilità di Governo in questo Parlamento - di aver sempre avuto la preoccupazione di dare assoluta priorità alle convocazioni del Parlamento, perché quello è il rapporto costitutivo in forza del quale un Ministro è tale. FI e AN).* Non sappiamo, al momento, quale sia il livello di questa riunione Italia-Qatar, ma credo che il Ministro potrebbe utilmente interrompere la sua riunione per venire in Parlamento. Visto che non siamo riusciti a ottenere questo risultato, forse è bene che siamo noi a sospendere questa seduta e a chiamare il Ministro perché non è possibile degradare la politica europea ad un livello tale che se ne parla come se non ci fossero in gioco questioni di valore, questioni politiche, questioni di linea di alto rilievo e di alto profilo. Qui stiamo umiliando un Senato che non lo merita perché nella discussione che avete ascoltato sono affiorate questioni di altissimo livello. C'è, per la verità, un'altra lettura possibile dell'assenza del ministro Bonino. Augusto Del Noce, mio grande maestro, insegnava che bisogna leggere i pieni ma anche i vuoti, le parole ma anche i silenzi, le presenze e anche le assenze: conoscendo un poco il ministro Bonino, onestamente alcune delle cose che ho visto e sentito in questa giornata credo che il Ministro non le avrebbe approvate; alcuni emendamenti sostenuti dal Governo dubito molto che il ministro Bonino avrebbe avuto la possibilità, possibilità, in coscienza, di sostenerli e di non dichiarare il consenso del Governo con le posizioni dell'opposizione. In molti casi sono passate infatti linee dirigiste, antiliberiste, posizioni le quali mostrano di avere un grande disprezzo delle regole fondamentali di funzionamento dell'Unione Europea. Se fosse vera la seconda interpretazione, crescerebbe la mia umana comprensione, ma il mio giudizio politico diventerebbe ancora più duro perché un Ministro deve venire in Parlamento a dire la posizione che in coscienza ritiene la migliore per il Paese e a dissociarsi, anche dalla sua maggioranza, se ritiene di doverlo fare. *(**Applausi dai È un segnale evidente dello scollamento e dell'agonia del Governo Prodi. Poniamo termine in fretta a questa agonia, il Paese non può permettersi una ancora più lunga agonia del Governo.

l'estro. Mi pare che oggi stiamo procedendo esattamente al contrario di come avremmo dovuto. Questa mattina ci siamo prodigati a spiegare al Ministro che, dopo quello che era successo ieri, forse sarebbe stato opportuno non venire qui e rinviare il dibattito su una materia così importante ad un chiarimento che doveva svolgersi all'interno del Consiglio dei ministri, ma nonostante i nostri appelli reiterati, la seduta è iniziata e siamo andati avanti. Nel pomeriggio ci troviamo nella situazione opposta, cioè il Ministro, che ha ottenuto dall'Aula di poter venire qui perché il provvedimento è importante, invece in Aula non ci viene. Vede, signor Presidente, ricordo un tempo nel quale in Senato in Senato non era consentito si svolgessero dibattiti se ai banchi del Governo non ci fosse almeno un Ministro. Era una tradizione del Senato molto rigorosa, che non valeva nell'altro ramo del Parlamento; lo ricorderanno i colleghi che sono stati Ministri in tempi non vicini a questo, ma ci voleva comunque la presenza di un Ministro. Oggi ci troviamo ad avere superato ogni limite: onorevole Sottosegretario, la ringrazio per quello che ha detto adesso, ma lei poco fa su un emendamento stampato ha detto a quest'Aula che aveva bisogno del tempo per leggerlo per esprimere un parere. Come è possibile che il rappresentante del Governo sullo stampato distribuito da ieri ha bisogno di tempo per leggerlo e dare il parere, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del lavoro che il Governo deve svolgere qui: possiamo aspettare che lei si legga gli emendamenti adesso per sapere qual è il parere del Governo? *(Applausi dai Gruppi* *FI e LNP)*. perché evidentemente non ha più pareri sulle cose di cui c'è bisogno nel Paese. Questo è il fotogramma di una tragedia italiana che continua ad andare in onda per la regia del professor Romano Prodi e di coloro che siedono nel Governo ma non vengono in Parlamento.

e attendere che il Ministro arrivi qui. Massimo rispetto per la Conferenza Italia-Qatar e massimo rispetto per il dibattito che questa

delle disposizioni del Consiglio ECOFIN relativamente alla politica economica e sociale dopo Lisbona. Non è possibile che il Governo non renda nota al Parlamento la sua posizione su questi temi. Il Governo può farlo, non è in agonia, anzi, deve farlo! Ci auguriamo che la ministro Bonino presti a questo dibattito perlomeno la stessa attenzione che presta alla trattativa sulle pensioni.

Da parte mia dichiaro che non accetteremo alcuna dilatazione dei tempi legata al fatto che oggi il Senato non è in grado di lavorare perché un Ministro non compie il proprio dovere!

chiedo che venga convocata il più urgentemente possibile una Conferenza dei Capigruppo per fare il punto della situazione. Almeno noi non intendiamo andare avanti a vista. Credo che abbiamo il diritto di sapere qual è il programma dei lavori del Senato, i quali non possono essere subordinati alla voglia di questo o di quel Ministro.

all'assenza del Ministro e quindi quella di ripristinare la condizione per la quale il Senato possa lavorare - è stato chiesto per primo dal senatore Salvi

deciso che la questione è rappresentata dal ministro Bonino perché la questione è il presidente del Consiglio Prodi. Evitiamo di credere che sia in gioco la questione del ministro Bonino!

A questo punto, è intervenuta la richiesta dei senatori della maggioranza e la Presidenza, ancor prima dell'intervento del presidente Castelli, ha aderito alla richiesta di sospensione. Ora vorrei capire se gli interventi dei senatori Salvi e Russo Spena abbiano

momento una Conferenza dei Capigruppo. Il fatto che lei stabilisca che, invece, si sospende la seduta nell'attesa del ministro Bonino instaura in quest'Aula un precedente che - a mio avviso - è contrario ad un'attenta lettura del Regolamento.

chiedendo se ancora questo Ministro facesse parte del Governo. Oggi pomeriggio il Ministro non c'è. non possiamo ignorare o far finta di ignorare che la polemica di ieri e l'assenza di oggi abbiano un significato politico. Non siamo disponibili, Presidente, ad attendere un'ora perché succeda qualcosa,

una richiesta corretta, perché questa umiliazione che viene nuovamente impressa all'Assemblea del Senato è davvero insopportabile. Non ci costringa, Presidente, a dover abbandonare l'Aula per l'ennesima volta in segno di protesta per questa continua rottura che c'è fra Governo e Parlamento.

discussione del disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007", avendo il ministro Bonino garantito per domani la sua presenza. del giorno, le ratifiche di Accordi internazionali e, come terzo punto, la discussione generale dei disegni di legge sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.